La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 4 ottobre 2007.

Come già previsto dall'ordine del giorno, seguiranno i disegni di legge sulla risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, sull'abolizione della pena di morte - per il quale è prevista la deliberazione a maggioranza assoluta e sull'introduzione del reato di tortura nel codice penale. Nella giornata di domani saranno discussi i disegni di legge recanti rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato, ove conclusi dalla Commissione bilancio. Per le votazioni finali è necessaria la presenza del numero legale. Gli altri disegni di legge che potranno essere esaminati nel corso di questa settimana sono quelli in materia di differimento termine delega professioni sanitarie e di sportello unico delle imprese, nonché ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione. Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 27 settembre, alle ore 14, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi (vale a dire dalle ore 14 in poi) gli onorevoli senatori; pertanto, la seduta antimeridiana del Senato si concluderà alle ore 13,45. Nel pomeriggio di giovedì 27 è previsto il *question time* con trasmissione diretta televisiva, rivolto al Ministro delle comunicazioni in tema di tutela dei minori nell'accesso ai sistemi informatici, e al Ministro dello sviluppo economico nelle seguenti materie: mafia-imprenditoria siciliana; fabbisogno energetico; andamento prezzi prodotti alimentari. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi nella mattina di martedì 2 ottobre per il seguito degli argomenti non conclusi. Il pomeriggio di martedì 2 sarà dedicato al seguito dell'esame del disegno di legge collegato sul riordino dei servizi pubblici locali, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 3 ottobre saranno discusse mozioni sul piano industriale di Alitalia, con particolare riguardo all'aeroporto di Malpensa. Nella stessa seduta avrà anche luogo l'esposizione economico-finanziaria del Ministro dell'economia e delle finanze. In relazione alla disponibilità del Ministro l'esposizione potrebbe essere anticipata alle ore 9.

e le altre mozioni eventualmente connesse sul vice ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Visco. Nella seduta antimeridiana di giovedì 4 ottobre sarà posta all'ordine del giorno la Nota di aggiornamento al DPEF, di imminente presentazione. L'organizzazione della discussione sarà definita dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre il Presidente renderà le proprie comunicazioni all'Assemblea sul contenuto del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, con conseguente inizio della sessione di bilancio. Seguirà il sindacato ispettivo. Queste sono le decisioni assunte questa mattina all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

Essendo state ritirate le proposte di risoluzione presentate, si intende così esaurita la discussione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge che viene sottoposto all'Assemblea nel testo già licenziato dalla Camera dei deputati, con votazione quasi unanime, contiene disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto tra datore di lavoro e lavoratori o prestatori d'opera. Tale dispositivo si pone l'obiettivo di eliminare la pratica molto diffusa delle false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell'assunzione, quando il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro. Ilcondizionamento prodotto da tale atto produce una pesante ricaduta sia sulla vita lavorativa, con la costante riduzione o rinuncia totale dei diritti in quanto lavoratrici o lavoratori, sia sulla propria vita affettiva, familiare e sociale. Il fenomeno di cui parliamo, molto diffuso, è difficilmente verificabile in quanto l'onere probatorio è a carico del lavoratore e in pochi casi si traduce in una prova scritta o testimoniale in grado di rendere nullo l'atto di cessazione del rapporto. È soprattutto in alcuni comparti produttivi, in particolare nelle piccole e medie imprese, dove l'estorsione delle finte dimissioni viene attuata in particolari condizioni, come la maternità, o per vantaggi fiscali, per sgravare l'assenza del lavoratore per eventi imprevisti, quali gli infortuni e la malattia. Se consideriamo che il lavoro è alla base di ogni progetto di vita, non deve quindi essere umiliato da pratiche vessatorie, specie in un quadro normativo che in questi casi risulta debole e inefficace. La stragrande maggioranza dei casi indagati dai sindacati riguarda soprattutto le donne e pertanto ci rendiamo conto dei grandi problemi sociali che possono nascere dall'esclusione delle donne da un progetto importante come la maternità, in un Paese dove le scelte procreative si rimandano sempre di più e dove la denatalità diventa un grande problema. È un Paese È un Paese che invecchia, il nostro; è un Paese che fa meno figli; dove una donna su cinque lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio, a causa di un *welfare* di sostegno estremamente debole. I dati dimostrano che laddove lavorano le donne si fanno più figli, le famiglie sono più ricche, crescono i consumi, cresce il prodotto interno lordo, cresce il Paese. E la società non può privarsi di queste risorse altamente scolarizzate, anche se meno retribuite a parità di mansioni. L'articolato che ci apprestiamo a votare avanza una proposta molto semplice, non onerosa, ma estremamente efficace: essa prevede l'obbligo, in caso di dimissioni volontarie, a pena di nullità, di procedere utilizzando dei moduli che presentano una numerazione alfanumerica progressiva, con una ridotta validità, per evitare contraffazioni e vincolare le dimissioni volontarie a meccanismi trasparenti. Essendo altresì stato presentato in Senato il disegno di legge Pisa, Mongiello ed altri, se ne propone l'assorbimento, essendo sostanzialmente analogo al disegno di legge n. 1695. A conclusione del mio intervento, voglio solo ricordare quanto sancito dall'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, oltre alla legge n. 300 del 1970, recante lo Statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, e l'insieme normativo delle misure a tutela della maternità e la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari, sulla cui efficacia si misura il benessere degli uomini e delle donne di questo Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra, anche dal numero degli iscritti a parlare, che questo disegno di legge stia passando in maniera assolutamente *soft*, in sordina, essendo per molti un disegno di legge che dovrebbe apparentemente tutelare le lavoratrici e i cosiddetti tartassati da coloro che si fanno firmare le cosiddette dimissioni in bianco. Credo invece che questa leggina vada introdotta, considerata e soppesata all'interno di un quadro più generale del mercato del lavoro, delle relazioni

alla possibilità di alleggerire e, a volte, di eliminare la rigidità del mercato del lavoro ci ha permesso un *trend* occupazionale in crescita costante e continua nel tempo.

incinte rappresentano, nella maggior parte dei casi o in alta percentuale, coloro che subiscono di più questo tipo di vessazione, cioè le dimissioni

ulteriormente i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. Qualcuno affermava che in alcune aree del Sud c'è una particolare propensione a questo tipo di vessazione, ma non è vero. Oggi non esiste più un'azienda che abbia la possibilità di farsi firmare in bianco le dimissioni da parte di un proprio lavoratore e, se qualche caso c'è, non credo che questo possa rappresentare lo strumento, per altro molto ideologico, da parte della maggioranza per percorrere ancora una strada di

irrigidito e per aver lasciato un segno negativo in quel mercato del lavoro che oggi poteva e può rappresentare la vera modernizzazione del Paese. Non credo che ci sarà un altro Governo, un'altra maggioranza, nella storia del nostro Paese, che possa, sotto la spinta di questa sinistra radicale e ideologica, permettersi un percorso

dovranno sopportare e subire e che irrigidirà ancora di più quel mercato del lavoro che invece dovrebbe essere il segno distintivo di ogni democrazia moderna e di ogni Nazione che voglia sviluppare il proprio progresso economico.

quasi sociale, diffuso soprattutto in un certa categoria di persone, gli imprenditori, la volontà di vessare la categoria dei lavoratori. Lo abbiamo visto

nulla: prima di uno o due anni, quando il Presidente della Repubblica ritirerà fuori quel discorso, non se ne parlerà più. Qui è la stessa cosa, nel senso che parliamo di un fenomeno che probabilmente - vista la frequenza con cui

e per forza su un modulo, stampato in maniera progressiva da enti pubblici, al di sopra di ogni sospetto (come possono essere i Comuni, l'Ispettorato del lavoro, gli uffici di collocamento e così via), così da evitare la possibilità che all'atto dell'assunzione vi sia una sorta di pre-licenziamento o di pre-dimissioni in bianco, cioè senza data.

accetterebbe mai una cosa del genere. Sarebbe impensabile tenere segreta una situazione simile; sarebbe impensabile che nell'azienda

la legalità - ripeto - è interpretata in maniera informale, per cui non ci si pone neppure il problema delle dimissioni preventive in bianco, per il semplice fatto che non ci si pone il problema delle assunzioni, nel senso che probabilmente la gente lavora in nero prima e dopo l'assunzione e il problema non esiste.

sindacal-comunista, anti-imprenditoriale, anti-aziendale, anti-industriale ed anti-tutto ciò che produce vera ricchezza.

in un Paese dove il problema è che si lavora poco in generale e che i pochi che hanno voglia di lavorare devono trascorrere la maggior parte del tempo a svolgere attività non lavorative per poter lavorare

i risultati si ottengono con leggi intelligenti, dove per legge intelligente si intende non una legge populista, ma una legge che conosce le regole del mercato e si comporta di conseguenza.

perché, paradossalmente, dando la possibilità di uscita dal mercato del lavoro si facilita l'ingresso in esso. Le aziende ampliano i propri organici andando a pescare nella parte non certa del fatturato, degli ordinativi e della clientela quando hanno la sicurezza che poi, nell'eventualità di una situazione peggiore rispetto alle previsioni, il carico di manodopera assunto in più possa essere in qualche modo liberato nel tempo. Il risultato finale è che la manodopera provvisoria diventa definitiva e che le aziende si consolidano su un livello di fatturato e di clientela più alto, come la legge 14 febbraio 2003,

Oggi non possono essere le aziende a pagare il 30, 40 o 50 per cento del periodo di maternità, perché non è giusto. Quello è un investimento collettivo che si deve pagare con il pubblico erario, con la pubblica fiscalità.

di questa situazione sull'azienda. Le aziende chiudono oppure non assumono donne giovani. Il problema è delle imprese che devono pensare soprattutto a salvaguardarsi o piuttosto dello Stato, incapace di intraprendere un minimo di legislazione di buonsenso e semplicemente di capire che il mercato esiste?

Volete avere un minimo di intelligenza per capire come funzionano le cose? Andiamo sulla strada da noi intrapresa che ci ha portato dal 10,5 al 7,5 per cento di disoccupazione e che voi, in questo anno, non avendo cambiato la legge n. 30, avete migliorato la situazione di un altro mezzo punto per cento. punto per cento. La situazione è questa. Per concludere, questa è la solita legge demagogica. Se dimostrate la buona volontà di accettare alcuni emendamenti, vuol dire che, perlomeno, con il beneficio del dubbio, la volontà buona nella direzione giusta c'era. Se li bocciate, è la solita legge

Signor Presidente, prendo la parola dopo interventi che condivido, come quelli svolti poc'anzi dai colleghi Piccone e Galli per enfatizzare la negatività di questo provvedimento, che non può essere in alcun modo sottovalutato. È ben vero che su di esso vi è stato un largo voto favorevole presso la Camera dei deputati, ma siamo in presenza della conferma dell'utilità del bicameralismo perché una lettura attenta di questo provvedimento solleva inevitabilmente le osservazioni critiche che coloro che mi hanno preceduto hanno già svolto. In modo particolare, vorrei ricordare il contesto nel quale si inserisce il provvedimento ha richiamato, poco fa, molto bene il collega Galli - quello di un mercato del lavoro straordinariamente rigido, nel quale in particolare la disciplina relativa alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro è stata considerata causa non secondaria di due connesse anomalie due connesse anomalie che hanno fatto del nostro mercato del lavoro quello che Marco Biagi definiva il peggiore nell'ambito dell'Unione Europea o, quanto meno, dell'Unione a 15. 15. Quello, cioè, caratterizzato contemporaneamente dai più bassi tassi di occupazione regolare - ed è questo un primato negativo che permane nonostante gli straordinari miglioramenti che si sono registrati nel corso dell'ultimo decennio a partire dal pacchetto Treu e, con una accelerazione significativa, successivamente alla legge Biagi successivamente alla legge Biagi - ai quali fa riscontro, peraltro, la più alta dimensione di lavoro sommerso. Concorrono a questa anomalia tutta italiana numerosi fattori, tra i quali certamente si deve annoverare l'altissimo costo indiretto del lavoro, quel 33 per cento di oneri previdenziali che colpevolmente questo Governo ha addirittura accresciuto rispetto al già altissimo livello del 32,7 La straordinaria onerosità del lavoro penalizza il salario netto e la propensione alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, ma in tale anomalia hanno un ruolo specifico anche il complesso di regole che riguardano il rapporto di lavoro e il complesso di oneri burocratici che caratterizzano l'accensione del rapporto di lavoro.

Bene, è proprio questa, tra l'altro, la platea di imprese nella quale forse si può ragionevolmente presupporre di riscontrare, seppure in misura assolutamente diversa da quella evocata dalla relatrice, la patologia delle dimissioni in bianco rese al momento dell'assunzione.

come ci segnala la Confartigianato, che insieme alla Confcommercio e alla Confindustria, ha rappresentato le ragioni per contestare questo provvedimento,

e quindi ha condannato il datore di lavoro a reintegrare in ogni caso il dipendente dimissionario nel posto di lavoro precedentemente occupato. Lo diceva benissimo il collega Piccone poco fa, si arriva anche alla prova della grafia, che consente di stabilire il momento dell'effettiva sottoscrizione delle dimissioni. Per non dire poi della particolare tutela che già oggi è disposta dall'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, a favore delle lavoratrici madri, e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 198

Ammettiamo per un attimo che la patologia sia così diffusamente presente, come voi dite e come a noi non risulta, questa per realizzarsi ha bisogno della forma scritta. allora, rendere comunque obbligatoria, nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore, la forma scritta? Cioè, ove le dimissioni non si realizzano con la forma scritta, caso che la giurisprudenza oggi costantemente riconosce (perché, per fortuna, vi è un principio pacificamente riconosciuto, quello della libertà di forma delle dimissioni e quindi dell'ammissibilità delle dimissioni per fatti concludenti), nel caso cioè in cui il dipendente sbatta la porta, non si ripresenti e quindi non ricorra alla forma scritta, e quindi non vi sia in alcun modo il dubbio che possa sussistere sotto quella forma scritta la patologia delle dimissioni

ma almeno non dovremmo costringere il datore di lavoro a rincorrere il lavoratore - che si è volontariamente allontanato e che ha mostrato un comportamento inequivocabile di rottura del rapporto di lavoro - con il modulo perché venga firmato e con ciò si chiuda consensualmente il rapporto contrattuale. Perché chiedete ciò? Il presidente Treu,

scritto». Senatore Treu, come deve leggersi questa legge e qual è la sua opinione? Occorre davvero la forma scritta? L'oggettività del testo impone la forma scritta? Se impone la forma scritta - come pensiamo - perché lo fa? Che cosa c'entra ciò con la patologia che avete richiamato all'origine del provvedimento? Perché si fonda tutta sull'uso della forma scritta? Perché chiedete questo? Temo che la risposta sia ancora una volta la lettura ideologica che prevalentemente date del rapporto di lavoro, l'idea che il rapporto di lavoro sia

Un'altra conseguenza di tale ossessione è quella per cui prevedete, con il provvedimento, di applicare il concetto di dimissioni anche a forme di lavoro autonomo, anche a quelle prestazioni che sono dedotte in contratto in relazione ad un risultato da produrre e per le quali le dimissioni non hanno senso e rappresentano una contraddizione in termini.

estendere a tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli di tipo autonomo, la la disciplina che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, nell'idea che le prestazioni di tipo indipendente siano anche esse un'anomalia, una patologia da ricondurre sempre e comunque alla subordinazione. Basti pensare che oggi le controversie che caratterizzano il rapporto di lavoro autonomo non rientrano nemmeno nella competenza del giudice del lavoro. Vostra intenzione, appunto, è quella di ricondurre tutto alla logica della subalternità del supposto contraente debole anche quando nei fatti, nella realtà fattuale, sono proprio norme come queste che rendono più debole il contraente, sono norme come queste che incoraggiano l'anomalia italiana per la quale pochi sono i rapporti di lavoro regolare, tanti sono i lavori sommersi: quella patologia tutta italiana che la legge Biagi ha cercato di rimuovere con alcuni parziali risultati, ma che voi continuamente, in controtendenza, cercate di contraddire con provvedimenti come questo.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

gli altri componenti della maggioranza, della Commissione in un altro, cioè se questo testo comporti o meno l'obbligatorietà della forma scritta nel caso di dimissioni volontarie. Gli emendamenti hanno lo scopo di chiarire che la forma scritta non è obbligatoria e che il ricorso a moduli a numerazione progressiva debba esservi soltanto nel caso in cui siano rassegnate per iscritto le dimissioni.

La seconda finalità, che alcuni emendamenti si propongono, è quella di non applicare queste disposizioni alle prestazioni di lavoro autonomo, per le quali il concetto di dimissioni non è proprio. Le prestazioni di lavoro autonomo sono prestazioni «a risultato», incluse quelle delle collaborazioni a progetto, che la legge Biagi ha definitivamente inquadrato nel lavoro indipendente, ancorché coordinato, cioè nel lavoro che si caratterizza per il risultato e non per la durata del rapporto.

queste posizioni di un adempimento in più che non ha senso, in quanto il rapporto è totalmente recepito nel contratto che viene stilato, sia esso a progetto o di altro tipo.

non modificano sostanzialmente il contenuto del provvedimento, mentre appare più importante in questo momento addivenire all'approvazione definitiva della legge. Per questo motivo, esprimo parere contrario.

Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

voteremo a favore di questi emendamenti. Riteniamo incredibile l'osservazione della collega Mongiello,

Insomma, senatrice Mongiello, volete o no la forma scritta obbligatoria nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore? Noi Noi leggiamo oggettivamente un testo che prevede l'obbligatorietà della forma scritta e ribadisco che tale obbligatorietà non ha nulla a che fare con la patologia che che avete richiamato, quella della dimissioni firmate in bianco dal lavoratore o, peggio ancora, dalla lavoratrice. Credo che, in realtà, voi seguiate un vostro percorso che, come ho detto, si ritrova anche nella riforma del processo del lavoro:

*pathos* un po' ossessivo e sinceramente incomprensibile, considerato che, invece, la discussione alla Camera ha avuto un andamento piano, conforme al carattere semplice della disposizione. Come ha detto poco fa la relatrice, non diciamo niente circa l'obbligatorietà della forma scritta delle dimissioni. Si prevede, piuttosto, che la lettera di dimissioni volontarie predisposta (la prassi che vogliamo combattere) è nulla se non è fatta nei modi

qui ci si occupa solo del caso in cui le dimissioni siano date con lettera preordinata. In generale, dunque, la forma resta libera, come è scritto in tutti i manuali e come da giurisprudenza. Stia pure tranquillo il senatore Sacconi

per lo meno tra le persone che abitano nei miei territori e che sono di quei territori: certo chi si chiama Brambilla, Bernasconi o Ravazzani certe cose non le fa. Vorrei invece chiedere al senatore Treu, ad esempio (vista l'origine della senatrice relatrice la Puglia, dove da qualche mese si scoprono laboratori clandestini dove danno 20.000 lire al mese a bambini di dieci anni, come si applicherà questa legge, oppure, per restare nella mia regione padana

che se il vice ministro Visco, che con la Guardia di finanza qualche problema ce l'ha, ma poi la sguinzaglia però solo dalle parti nostre (non solo dalle nostre parti geografiche, ma dalle nostre parti etniche, perché in Lombardia controllano solo

il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.103, che mi dà l'occasione per confermare al senatore Treu una lettura, quella che facciamo della lettera oggettiva del provvedimento, ricordandogli che essa è condivisa da tutte le associazioni dei datori di lavoro italiane, che hanno espresso le critiche che oggi qui abbiamo manifestato.

In primo luogo, vorrei vedere qual è quel giudice del lavoro che di fronte a un lavoratore che dichiara che la sua lettera di dimissioni è stata postdatata e gli è stata estorta con metodi surrettizi non gli dia ragione; credo non ce ne sia nemmeno uno in tutta Italia. Quindi, facciamo una legge per combattere il nulla. In secondo luogo (mi rivolgo un po' a tutti), siamo accusati in questo momento dalla cosiddetta antipolitica che sta prendendo piede nel Paese

si intende costruire un modulo che deve essere realizzato secondo le direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Quindi, i due Ministri si trovano per stabilire che modulo devono costruire, poi entro tre mesi emanano la norma per cui viene definito il modulo; anzi, il modulo deve avere un codice alfanumerico progressivo di identificazione, deve avere la data di emissione, nonché spazi da compilare a cura del firmatario, in cui gli chiederanno chissà che cosa, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni alto elemento utile.

e saranno altre spese per lo Stato e per il Governo. Noi stiamo legiferando su questo, colleghi; stiamo legiferando su questo. Allora, quasi quasi mi iscrivo al partito di Grillo, perché perché credo veramente che quando lui critica la classe politica che perde tempo a fare queste cose abbia mille e una ragioni.

all'altro aspetto del provvedimento in esame, quello per il quale si vuole estendere il concetto delle dimissioni volontarie alle prestazioni di lavoro indipendente, che sono prestazioni a risultato e non di durata. Come tali esse sono concettualmente incompatibili, a meno che non si voglia - come si vuole con il provvedimento- ricondurre o cercare di ricondurre quanto più anche la disciplina del lavoro autonomo alle caratteristiche del lavoro subordinato. Ricordo che la legge Biagi - insisto - ha assimilato anche le collaborazioni a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative, alle prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro indipendente

Senatore Castelli, se lei è d'accordo, poiché il quesito che lei ha posto esula non solo dall'emendamento che stiamo per votare, ma anche dai successivi,

sia particolarmente colpevole e sarebbe almeno opportuno limitarla solo al provvedimento in esame, senza dare ad essa una valenza più generale. Anche per questa votazione chiedo l'uso del supporto elettronico.

a contrastare l'allargamento del deprecabile uso delle dimissioni in bianco. Ho constatato che, a parte qualche isolata voce, l'argomento ha registrato massima convergenza sia nelle sedi di esame che nella discussione alla Camera dai Gruppi politici di maggioranza, nonché dal Governo che valuta con favore tale disciplina. Adduco tale inconsueto accordo alla comune consapevolezza di arginare la prassi ai limiti della legalità di richiedere ai lavoratori dimissioni firmate in bianco contestualmente all'assunzione. Questi sono atti riprovevoli ed inaccettabili perpetrati ai danni dei lavoratori ed ancora più delle lavoratrici, che costituiscono un vecchio retaggio discriminatorio di inciviltà sociale non più tollerabile nel terzo millennio. Ecco perché ribadisco, in uno con il mio partito, l'urgenza di un intervento legislativo risolutivo ed esprimo piena adesione al progetto qui all' esame, di cui è auspicabile una sollecita approvazione. Anzi, sostengo che il disegno di legge in titolo andrebbe perfezionato con l'adozione di una disciplina inasprita, che in maniera decisa ed efficace faccia cessare la pretesa di chiedere firme su un foglio bianco per poi avvalersene a piacimento in un momento successivo. Devo altresì evidenziare a voi colleghi che il fenomeno è riscontrabile nel Mezzogiorno con frequenza ancor più preoccupante e pertanto va immediatamente e drasticamente impedito, se vogliamo continuare a sostenere politiche per il Sud e per il Mezzogiorno d'Italia. Aggiungo poi il monito di non fermarsi a misure isolate, ma dare seguito ad interventi legislativi congeniati al fine di superare le varie disparità di trattamento che penalizzano ancora i lavoratori e assicurare nell'ambito del diritto del lavoro adeguati livelli di tutela. In conclusione, constatando la positività e la bontà dell'iniziativa legislativa, esprimo voto positivo all'Atto Senato in esame.

ha un grande obiettivo e - anche il senatore Sacconi era d'accordo - ha un grande effetto, quello di opporsi all'illegalità e all'ingiustizia, che penso dovrebbe essere un valore condiviso, che nel nostro Paese colpisce i soggetti più deboli. Parlo dei tanti lavoratori privi di un vero e proprio potere contrattuale, per esempio parlo di quelli che hanno condizioni di sicurezza sul lavoro molto lacunose. In quest'Aula si è parlato tante volte delle morti bianche, sono stati 1.600 i lavoratori deceduti l'anno scorso, o i soggetti privi addirittura di qualsiasi contratto, come per esempio le nuove schiavitù create dalla diffusione del caporalato in agricoltura e nell'edilizia, si trovano anche sui viali romani, non solo nel Sud dell'Italia, e penso anche al Nord. Le lavoratrici e i lavoratori si trovano di fronte ad un *diktat*: "prendere o lasciare", che è lo stesso del caso di cui trattiamo oggi, quello cioè delle dimissioni in bianco. Si tratta di un fenomeno ricattatorio, sintomo dell'illegalità diffusa che si realizza quando alcuni datori di lavoro al momento dell'assunzione come diceva prima la collega Mongiello, il lavoratore è più debole - fanno firmare alle lavoratrici una preventiva lettera di dimissioni con data in bianco, che può essere usata a totale discrezione del datore di lavoro. È una spada di Damocle che pende sulla testa di tanti lavoratori, e soprattutto lavoratrici, utilizzata per interrompere un rapporto di lavoro in caso di maternità, di infortunio o di malattia. È una pratica molto diffusa che sgrava l'impresa dai pagamenti del periodo di assenza ed aumenta la precarietà del lavoro,

Soprattutto, però, le dimissioni in bianco precludono alla lavoratrice e al lavoratore di percepire l'indennità di disoccupazione. Si tratta di un effetto economico devastante: non si guadagna e non si mangia. Il funzionamento difensivo previsto da questo provvedimento è elementare. La validità delle dimissioni volontarie non è burocratica, è molto semplice: è vincolata all'utilizzo da parte dei lavoratori di moduli predisposti, usufruibili solo attraverso gli uffici competenti, datati e contrassegnati da codici progressivi, con una validità di 15 giorni dalla data di emissione. al punto che se tutte le pratiche burocratiche del nostro Paese fossero semplici come l'utilizzo di questo modulo, saremmo un pezzo avanti! Una norma semplice, dunque, concreta e di buonsenso, fortemente condivisa alla Camera che rappresenta una norma di civiltà e che sana una pratica odiosa e purtroppo molto diffusa. Non solo. Si tratta di una norma preventiva rispetto ad ipotetiche denunce ed azioni giudiziarie - e quindi non onerosa - e, soprattutto, rispetto al sorgere del problema. Infatti, se è vero che ci sono altre leggi, sono tutte *ex post*. anziché ricorrere a divieti e multe punitive, adotta una semplice pratica di trasparenza e di risoluzione pacifica di possibili problemi: un esempio di quel diritto mite che invochiamo sempre in quest'Aula e che va nel senso del rispetto della Costituzione. Questo provvedimento, assolutamente non oneroso, tende ad un relativo riequilibrio delle posizioni nel rapporto di lavoro, sottraendo le lavoratrici e i lavoratori a quello che si può chiamare ricatto, abuso di potere, piccola furbizia che lede la dignità del lavoro e, soprattutto, costituisce un attacco alle condizioni materiali di vita, perché di questo si sta trattando. La figura più colpita è quella delle lavoratrici che scelgono di diventare madri. Già la precarietà colpisce più le donne che gli uomini (a fronte del 63 per cento di donne precarie, vi è solo il 37 per cento di uomini); in caso di maternità poi, con il meccanismo vigente di dimissioni in bianco, le donne vengono allontanate dal lavoro e la loro scelta è

si colpevolizzano le giovani donne, imputando loro la denatalità dell'Italia, come qualcuno tra voi ha detto. Inoltre, non solo mancano le strutture sociali di conciliazione, e manca la condivisione tra lavoro e accudimento dei figli all'interno della famiglia con i *partner*, ma la donna che sceglie la maternità e che ha bisogno del suo lavoro per mantenere il figlio viene punita con un licenziamento mascherato da dimissioni. Ma non è un grave controsenso?

sono casi veri. I dati forniti dall'Ufficio vertenze della CGIL riferiscono di 1.800 le donne che, ogni anno, chiedono assistenza legale, cioè un procedimento burocratico formale, per estorsione di finte dimissioni volontarie. Ciò avviene quando il fatto è già avvenuto e il posto già perso. Si stima, inoltre, che solo una lavoratrice su dieci ricorra al giudice del lavoro.

sia dal punto di vista contrattuale (e mi riferisco alla condizione concreta dell'esistenza delle donne legata alla necessità di un salario per vivere) sia da quello simbolico in quanto le donne, con questa legge, saranno più padrone della loro vita.

Chi si oppone a questo provvedimento deve spiegare perché vuole mantenere una situazione di illegalità, che non solo minaccia le regole della competitività (e questo dovrebbe interessarvi perché tra le aziende che assumono regolarmente e quelle che utilizzano lo strumento illegale delle dimissioni in bianco esiste una ma, soprattutto, mantiene lavoratrici e lavoratori in una situazione di ricatto perpetuo. Noi abbiamo presentato questo disegno di legge l'8 marzo

Colleghe, colleghi, signor Presidente, questo è un voto che dobbiamo alle donne, alle loro scelte, ai loro percorsi, alla fatica in più delle loro vite: la politica e il Parlamento hanno un'occasione per non deluderle. Mi auguro che il Senato approvi questo provvedimento. Sinistra Democratica, che lo ha proposto alla Camera e al Senato raccogliendo l'adesione di tante e tanti parlamentari, lo farà convintamente.

senza possibilità di emendamenti, quindi introducendo le dimissioni scritte anche laddove non sono previste e laddove la fattispecie dell'illegalità, del reato o dell'azione illegittima che dir si voglia, non erano fisicamente possibili, dimostra che stiamo parlando di altra

tanto che, nel mondo, i Paesi in cui la classe operaia sta meglio sono i Paesi liberisti, a libero mercato, dove si applicano i princìpi della concorrenza e della flessibilità del lavoro. Mi sembra che gli esempi, invece, di economia socialista reale siano proprio quelli in cui non certo i burocrati del partito che hanno la dacia nella foresta per l'inverno e la dacia in Crimea per l'estate, ma proprio la povera gente effettivamente se la passa peggio. Quindi, dovrebbe bastare questo per farvi cambiare idea, però apprezzo le persone di fede. Se dunque anche di fronte

per questioni democratiche ovviamente perché devono piangere i ricchi, ma evidentemente anche tutti gli altri. Infatti, siete riusciti contemporaneamente ad abbassare gli stipendi delle classi più deboli del Paese, ad aumentare le tasse agli imprenditori, ad aumentare gli studi di settore e di settore e gli obblighi burocratici delle aziende e adesso aumenterete anche la tassazione sulla rendita finanziaria, facendo dell'Italia l'unico Paese al mondo che non fa scelte, che non decide di privilegiare il lavoro o la rendita: ammazzate tutti e due e fine delle trasmissioni, senza così

a meno che volevate - ma non è questo il caso - colpire quelle sacche di irregolarità e di illegittimità che esistono anche nelle mie zone, ma che non sono certo perpetrate e vissute dalle persone delle mie zone. Anche in questo lo Stato ha una doppia velocità oltre che una doppia vista.

nel tragitto dalla caserma alla fabbrica del signor Brambilla passa davanti a 20 venditori ambulanti abusivi, dieci magazzini sotterranei di cinesi, dieci laboratori abusivi di cinesi

è che ormai il Paese è spaccato in due, non solo come storicamente ovvio anche dal mio punto di vista. Ormai è spaccato in due un'altra volta. C'è un Paese della legalità,

oltre ai milioni di italiani che avevamo già. Ciò posto, la parte che appartiene al Paese legale è sempre più piccola, ha un peso sempre più grande, e voi continuate a martellare questa piccola parte che mantiene una parte sempre più grande e che vive nell'assoluta illegalità.

gli 800 collaboratori in nero erano tutti del centro-destra? Mi sembra che con la conformazione di Camera e Senato in questa legislatura, se erano 800 almeno una bella fetta doveva

Governo e di una maggioranza che esprime personaggi di un certo tipo. Pensiamo a Ferrero, che non si preoccupa degli italiani o dei piemontesi, visto che lui è piemontese, ma incita gli immigrati ad andare in piazza per i diritti a Mastella, che manda via i magistrati scomodi e che fa arrestare per direttissima uno che gli ha tagliato la cima della barca (forse perché dormiva e rischiava di trovarsi in mezzo al mare senza saperlo), Visco che viene qui ad aumentare gli studi di settore e che, come si diceva sui giornali (oltre che dover dare un'occhiata alla sua Puglia), ha la villa abusiva, o parzialmente abusiva, a Pantelleria ed ha applicato il condono Berlusconi,

una volta che una persona non prende più uno stipendio dallo Stato ma la pensione, cosa cambia per il pubblico Erario? La differenza è che invece di tre stipendi dopo ne avremo quattro. Con questa gente complimenti e auguri al Paese.

gli stessi appartenenti alle forze che hanno espresso un parere favorevole alla Camera qui esprimono un parere contrario. vuol dire che o i vostri colleghi della Camera hanno l'anello al naso, per così dire, o c'è proprio un po' di schizofrenia, oppure

Anziché discutere nel merito del provvedimento, si portano altre argomentazioni. Infatti, non ho sentito nessun senatore dell'opposizione sostenere che chiedere le dimissioni in bianco ad un lavoratore o ad una lavoratrice sia un comportamento accettabile; anzi, è un comportamento assolutamente criticabile che va condannato e combattuto. Allora, non vi capisco più, perché questo provvedimento dice unicamente questo. Siamo di fronte ad un fenomeno che vede sempre più aumentare il ricorso da parte dei datori di lavoro

una situazione insostenibile di inciviltà. Questo è un disegno di legge molto scarno che risponde ad una norma di civiltà

È quantomeno dimostrabile, per la sequenza alfanumerica dei singoli provvedimenti,

su altre questioni, si parli d'altro. Parliamo nel merito. Nel merito vi ho sentiti tutti dire che, se un datore di lavoro chiede ad un lavoratore o ad una lavoratrice di firmare una lettera di dimissioni in bianco, quel datore di lavoro è condannabile. Bene, se così è,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che questa Aula si appresta a licenziare si riferisce, evidentemente, al fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, dell'assunzione si chiede alla lavoratrice ed al lavoratore la sottoscrizione di una lettera di licenziamento volontario in bianco, una lettera che verrà messa in un cassetto, pronta per essere usata quando successivamente converrà al datore di lavoro. Tuttavia, come spesso accade in questa legislatura, le lodevoli intenzioni del legislatore vengono poi afflitte e appesantite da un clima ideologico che ne svilisce la definizione normativa. Capita così che interventi mirati verso la maggiore efficacia di norme già esistenti devono cedere il passo a nuove leggi che, nel migliore dei casi, non risolvono i problemi e si risolvono in un inutile appesantimento degli oneri burocratici di cui, certo, il mondo del lavoro serio e operoso non ha bisogno. Rispetto al fenomeno che questo disegno di legge intende principalmente colpire, ossia la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, che, come si legge nella relazione introduttiva, riguarda prevalentemente le donne lavorataci, si ritiene non sia ravvisabile nessuna reale necessità di un provvedimento di legge specifico, perché esiste già, nel nostro ordinamento, una normativa e una tutela giurisdizionale adeguata contro questi abusi. Dal punto di vista normativo, infatti, le ipotesi delle dimissioni in bianco delle lavoratrici, in caso di maternità o di matrimonio, risultano regolamentate nel nostro ordinamento. dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento dev'essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006 stabilisce la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (purché segua la celebrazione) ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla direzione provinciale del lavoro. Infine, è noto come la giurisprudenza sia particolarmente attenta a tutelare i lavoratori in fattispecie siffatte, ritenendo nulli gli atti di recesso così formulati e sanzionando il datore di lavoro con la reintegrazione del dipendente dimissionario nel posto di lavoro precedentemente occupato. Ciò premesso, volendo tralasciare ogni valutazione circa la necessità di un intervento legislativo in materia, resta il fatto che l'attuale disegno di legge, per la sua formulazione, finisce con l'introdurre un meccanismo che complica e appesantisce la gestione del rapporto di lavoro e, allo stesso tempo, lascia il dubbio interpretativo circa l'effettiva portata della disposizione. Invece di soluzioni eque e concordate tra tutti i soggetti interessati e razionali dal punto di vista dell'efficacia comunicativa, ci si è voluto affidare a soluzioni cartacee ed arcaiche che peraltro creano problemi nuovi e non certo privi di rilevanza. Basti pensare solo, per fare un esempio, all'abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore e alla sua eventuale inerzia nel comunicare per iscritto le proprie dimissioni con la modulistica che qui viene richiesta. Ci si troverebbe di fronte ad un conseguente stato di incertezza sulla esistenza stessa del rapporto di lavoro ed obbligherebbe l'impresa ad attivare le procedure di licenziamento con perdite di tempo ed ulteriori danni economici. E l'abbandono del posto di lavoro non sembra certo un'ipotesi né insolita né infrequente nella prassi, specie con riguardo ai lavoratori migranti. Appare inoltre inaccettabile l'estensione del campo di applicazione del provvedimento in esame anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alle prestazioni occasionali di collaborazione, ai contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. Tale previsione normativa finirebbe con il comportare l'estensione al rapporto di lavoro autonomo di norme ed istituti, come quello delle dimissioni, che da sempre afferiscono al solo rapporto di lavoro subordinato. Tale estensione del campo di applicazione, che sembra sottendere una più generale ed inaccettabile intenzione del legislatore di eliminare dall'ordinamento giuridico la categoria del lavoro autonomo, è assolutamente da evitare anche sotto il profilo sistematico. Basti pensare ad esempio che, fatta l'eccezione dei soli rapporti di parasubordinazione, le controversie concernenti gli altri rapporti di lavoro autonomo richiamati dalla norma di cui trattasi non rientrano neppure nella competenza del giudice del lavoro. Quando ci troviamo di fronte a certi provvedimenti si è soliti dire che è necessario riequilibrare il differenziale di potere contrattuale che esiste tra l'imprenditore e il lavoratore. A mio avviso si è persa ancora una volta l'occasione per dare un segnale politico equilibrato. L'assoluta chiusura del Governo e della maggioranza a qualsiasi costruttiva modifica ci rende sereni nell'esprimere il nostro voto contrario a questo assurdo provvedimento.

veniamo sottoposti spesso a manifestazioni di cultura razzista? Lo sottolineo: razzista. È indispensabile che dobbiamo esserne in qualche modo complici? Penso che questo sia un problema. Non è la prima volta: è capitato ancora quest'oggi più di una volta. Domando se c'è un codice di comportamento che dobbiamo tenere. Comincio il mio intervento nel merito col dire che credo che ciascuno abbia diritto alle proprie retoriche e alla fissità di certi propri riferimenti, ma penso anche che quando si ragiona su una cosa, un limite vada trovato nel senso di realtà. Il senso di realtà che la Camera dei deputati, di fronte a questo provvedimento, in qualche modo ha trovato e che oggi invece mi sembra non ci sia stato nel dibattito. chiamare in campo le sciagure derivanti da tutta questa rigidità o l'appesantimento di un provvedimento burocratico che questa norma potrebbe comportare, mi sembra eccessivo. Stiamo parlando di una tutela minima, semplice. Tra i contraenti non c'è una parità: ci sono forze e poteri diversi. Queste forze e poteri diversi vanno in qualche modo equilibrati. Penso che questa sia una buona legge perché cerca un riequilibrio, cerca di tutelare di più la parte che in quel momento è più debole, la parte che ha meno possibilità e meno garanzie. Oggi comunque è una buona giornata per l'autodeterminazione delle donne, perché passerà questa legge e il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea convintamente la voterà. Una legge semplice, è stato detto: infatti. è composta di un solo articolo chiarissimo, che può capire chiunque. Si racchiude in un solo preciso articolo una misura per contrastare la pratica delle dimissioni estorte al momento dell'assunzione, soprattutto a lavoratrici, ma anche a lavoratori. Una pratica, è stato detto, illegale, che colpisce soprattutto le donne e riguarda una cultura di impresa, della piccola e media impresa in particolare, che considera più oneroso, meno conveniente assumere una donna, per i costi connessi alla possibile gravidanza e alla maternità e - aggiungo - alle tutele che da lunghi anni in questo Paese sono garantite per la maternità, come Dopo che questo testo sarà stato licenziato dal Parlamento, la validità delle dimissioni volontarie del prestatore d'opera sarà condizionata alla loro formulazione apposta su un apposito modulo, numerato e datato, non consentendo quindi di estorcerle al momento dell'assunzione. Semplice ed efficace. Semplice come può esserlo può esserlo una norma che nasce da una internità al mondo del lavoro e da una conoscenza, anche pratica, dei suoi meccanismi, tanto da poterne impiegare qualcuno a favore della parte più debole: perché, come dicevo prima (non si deve dimenticarlo mai), tra il lavoratore e la lavoratrice non c'è un rapporto paritario, c'è una asimmetria forte, in cui la parte datoriale, il padrone, è più forte e compito dello Stato - e con questa legge un pezzo di questo lavoro si fa - penso sia esattamente quello di interporsi tra le parti, equilibrando le forze

perché, nell'assumere forzatamente, necessariamente, un punto di vista sessuato, che muove dal differente collocarsi nel mercato del lavoro dei soggetti, propone una soluzione che è di tutela per uomini e donne, ma per queste ultime amplia amplia l'orizzonte della libertà, della propria autonomia e quindi, in ultima istanza, della propria possibilità di un'autodeterminazione. Il fenomeno delle dimissioni in bianco è per sua natura difficile da misurare, per le difficoltà nel farlo emergere e nell'analizzarne le cause, ma i dati e le ricerche ci

a muovere il datore di lavoro a questa pratica: ci sono i periodi di infortunio, le malattie lunghe; c'è la richiesta di applicazione della legge n. 104 del 1992, quando si ha un parente gravemente handicappato, che diventa già motivo per cui la lavoratrice o il lavoratore è pesante, costa troppo. Si tratta, cioè, di tutte quelle condizioni che rendono il lavoro, considerato come pura merce, più costoso, meno produttivo, e per abbatterne i costi e aumentare il profitto si impone questa pratica brutale. È una cultura diffusa, questa, che trova nella precarizzazione del lavoro - quella che viene chiamata flessibilità postfordista

e di dissolvimento del legame sociale non si può più ormai non tener conto, affrontando tali questioni in modo coraggioso, più coraggioso di quanto non si è fatto fino adesso. La legge non affronta questa problematica, ma è un utile passo per affermare la dignità del lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori. Molti sono gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro: la prima è l'iniqua divisione del lavoro di cura, ma poi c'è la carenza dei servizi di cura all'infanzia quanto ai malati anziani, il differenziale salariale che permane forte tra uomini e donne e poi quel rischio di povertà connesso al fatto che le pensioni delle donne sono più basse. Su questi motivi è urgente intervenire. esame non sta a quel livello lì, ma di fronte a noi si apre un periodo di discussione sulla finanziaria in cui vogliamo sperare e vogliamo lavorare perché questi aspetti vengano affrontati. Per tali motivi voteremo convintamente a favore di questa legge. Ho detto però all'inizio del mio intervento che c'è più di un motivo oggi per essere in qualche modo contente perché si fa un passo nel senso dell'autodeterminazione delle donne: il secondo motivo lo dico alla fine ma comunque non posso esimermi dal rilevarlo, ed è che oggi su tutti i giornali si parla della sentenza del tribunale di Cagliari

contente perché riapre una discussione, perché rimette quella legge, che si è persa nei cieli assoluti dell'ideologia autoritaria e repressiva, con i piedi per terra, la rimette in un posto dove i soggetti reali, donne e uomini, coppie, madri, possono discutere e possono scegliere.

condivide quanto già fatto dai propri colleghi della Camera. Riteniamo che questo provvedimento

dalle questioni che di fatto si discutono, si elaborano e si votano. Ritengo che contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che pure esiste, sia un fatto di civiltà, come dicevo prima. Credo che non ci possa essere un riferimento di carattere ideologico-partitico a questo modo di procedere:

scrive una lettera, in questo caso su un modulo che deve effettivamente essere a disposizione in modo che non si crei assolutamente alcun problema. Ora, se vogliamo caricare di problemi questo modulo, credo che stiamo parlando di altro. quindi apprezzato molto, anche rileggendoli, gli interventi, le dichiarazioni di voto della stragrande maggioranza dei colleghi dell'opposizione della Camera dei deputati, dove tutti hanno votato a favore di questo provvedimento.

acquistino efficacia decorsi 15 giorni dall'effettiva disponibilità dei moduli di cui all'articolo 1, comma 1, nella forma prevista dal successivo comma 5.

che si manifestano in maniera anche prepotente, soprattutto nel profondo Sud, nella criminalità organizzata, alle imprese. Sono due cose diverse, completamente diverse. L'imprenditore al Sud fa l'imprenditore e, salvo una piccolissima fetta collusa, sta sul mercato e lavora mercato e lavora in maniera eguale a quelli del Nord; anzi, probabilmente in un regime di selettività maggiore, in un regime di infrastrutture e di servizi minori, quindi con più difficoltà. L'imprenditore al Sud,

sulla quale probabilmente c'è anche da andare a verificare dove, come e in che quantità; si tratta veramente di una patologia. Questa precisazione non polemica, siccome ogni volta si accosta l'imprenditoria del Sud con l'illegalità, credo sia doverosa. Invece nel provvedimento (che è l'aspetto più importante), proprio a fronte di questa patologia (stiamo parlando di dimissioni per iscritto in bianco, presunte, fenomeno che a noi non risulta essere così diffuso), si intende colpire tutto il resto del mondo del lavoro, tutto l'apparato, l'apparato, che in qualche modo si vedrà costretto non più a seguire i canoni classici seguiti finora, in considerazione del fatto che comunque esiste una giurisprudenza che acclara come il recesso dal contratto di lavoro in questa maniera, per difetto di causa, viene ritenuto nullo e quasi sempre - esistono le statistiche - i giudici del lavoro, molto attenti, reintegrano il lavoratore nel posto di lavoro. Allora, non potendo o non sapendo colpire questa patologia, cosa facciamo? Estendiamo questo vincolo a tutti. Provo a farvi pensare che cosa succede nel caso un lavoratore e accade spesso - sbatte la porta perché è in conflitto con il proprio datore di lavoro, soprattutto nelle piccole aziende, e non firma alcun modulo. Vorrei capire se in quel caso il datore di lavoro da vittima deve passare ad essere "carnefice" e rincorrere il lavoratore, perché in quel caso dovrebbe dimostrare, attraverso tutta una serie di situazioni lunghe e difficoltose (voi lo sapete bene), che quel lavoratore si è dimesso dal posto di lavoro se si rifiuta di firmare il modulo. Credo che questa sia invece di fatto l'anomalia più grande. Ma non è la sola. Caro collega Tibaldi, ti preoccupavi di sapere se il collega Castelli avesse mai lavorato: io provo a indovinare che, da sindacalista, avrai lavorato probabilmente meno tu di lui; non conosco l'età e i lavori che fate, ma ti assicuro che di sindacalisti e di tuoi colleghi distaccati e in missione ne ho visti tanti e pochi ne ho visti a lavorare. Anche Anche se in difformità con i colleghi della Camera dei deputati, che in sede di dibattito probabilmente avranno approfondito in maniera diversa il provvedimento, ti meravigli tu, caro collega,

di fingersi non eterosessuale, altrimenti non si riesce ad avere le introduzioni giuste, perché ormai è all'ordine del giorno. La cosa più grave (io almeno credo sia la più grave) è il fatto di estendere questa normativa ai lavoratori autonomi, ai lavoratori a progetto. Noi vogliamo regolamentare attraverso un modulo che un imprenditore di se stesso deve dimettersi da se stesso! Redige un contratto con l'azienda, un contratto che è un progetto, che ha un obiettivo, che ha una finalità, che viene retribuito a seconda del raggiungimento di questo obiettivo, e si dimette: da che cosa? La verità è un'altra; la verità è che in questo modo,

Nel momento in cui tutto il mondo si interroga e diversi Paesi procedono ad estendere la flessibilità sul lavoro anche in uscita, seppur accompagnata da grandi ammortizzatori, noi addirittura vogliamo combattere quell'unica conquista fatta, che con dati alla mano

aveva potere di veto sulla collocazione in Borsa di una delle aziende più floride e più sane, forse una delle poche aziende sulle quali possiamo vantarci di avere la

molto più di quello che pensate di fare voi con i lavoratori. Se oggi il lavoratore comincia ad avere un appesantimento del rapporto con il datore di lavoro lo deve proprio a questo tipo di atteggiamento. Noi abbiamo invece la necessità di difendere la classe imprenditoriale piccola e grande, insieme con i lavoratori seri, quelli che lavorano e non quelli tutelati inopportunamente, quelli che stanno sul posto di lavoro cercando di fare il proprio dovere, avendo come faro principale la meritocrazia e il senso del dovere. Dobbiamo difendere gli uni e gli altri contro questa visione marxista, ottusa e retrograda che ci farà tornare ad un mondo del lavoro dell'800.

Signor Presidente, anch'io voglio sottolineare che il disegno di legge in discussione è esclusivamente finalizzato all'esigenza di contrastare una prassi molto diffusa e che determina gravi violazioni dei diritti dei lavoratori.

La prassi in base alla quale il datore di lavoro può firmare alla lavoratrice o al lavoratore una lettera di dimissioni con data in bianco, prima - e questo è un altro punto importante - della stipula del contratto di lavoro, di fatto aggira l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 e colpisce, com'è stato detto da più interventi, soprattutto le lavoratrici.

la possibilità, in caso di dimissioni volontarie, di procedere utilizzando dei moduli specifici rappresenta, per il lavoratore e la lavoratrice, uno strumento che può garantire l'effettiva volontarietà delle dimissioni, quindi uno strumento di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, e non un vincolo per i lavoratori e per le aziende. Si è molto discusso attorno a questo problema, circa la volontarietà o meno di quest'obbligo. È del tutto evidente - insisto - che non c'è nessun obbligo, non c'è nessun vincolo: si tratta di una possibilità che viene consegnata ai lavoratori e alle lavoratrici per tutelarsi. È risaputo, e chi ha lavorato in fabbrica lo sa forse più di altri, che il lavoratore non è obbligato, se vuole andarsene, se vuole licenziarsi, a sottoscrivere sempre le dimissioni. Il lavoratore può benissimo non farlo,

Presidente, penso che si possa accogliere la richiesta del senatore Tofani come ordine del giorno, se egli intende formalizzarlo.

senatore Sacconi

Ricordo altresì che per la votazione del disegno di legge è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato, ovvero 162 senatori. Il relatore,

Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, signor Presidente, abbiamo già discusso ampiamente e con animo unitario questo importantissimo cambiamento della Costituzione che elimina, anche per i codici militari in caso di guerra, la possibilità della pena di morte.

Vorrei ricordare a tutte le colleghe e i colleghi un'altra pena di morte, che non viene mai nominata, ma che pena di morte è: mi riferisco alle famose esecuzioni mirate di Israele nei Territori palestinesi occupati.

la storia del nostro Paese. Spesso si abusa di quest'espressione, ma non è questo il caso. Con l'approvazione in seconda lettura, e quindi in via definitiva, di questa modifica costituzionale, l'Italia diventa un Paese totalmente abolizionista e si completa un cammino iniziato nel 1889, con la promulgazione del codice Zanardelli, successivamente riproposto con la Costituzione repubblicana e con l'articolo 27. In quell'articolo il ricorso alla pena capitale era ed è escluso ad eccezione dei casi previsti dalle leggi militari di guerra: con l'odierno provvedimento cancelliamo anche quell'eccezione. Già il 13 ottobre del 1994 era stata promulgata la legge n. 589 che aveva cancellato la pena di morte dal codice penale militare di guerra, ma il quarto comma della Costituzione rendeva possibile in un futuro la sua reintroduzione. Cancellando oggi tale previsione dalla nostra Costituzione trasformiamo il nostro Paese in un Paese totalmente abolizionista. Da

definire finalmente una moratoria universale delle esecuzioni capitali di cui il nostro Paese è primo e diretto protagonista.

una posizione comune di sostegno a questa iniziativa italiana e su tale posizione si stanno allineando diversi Paesi. È un cammino lungo quello che si è

il Gruppo di Sinistra Democratica vota convintamente a favore di questa modifica costituzionale per di dare, con il voto di oggi, un contributo fondamentale e per compiere un passo avanti rispetto alla civiltà giuridica del nostro Paese.

che l'ultima condanna a morte comminata in Italia fu eseguita il 4 marzo 1947, cioè 60 anni e mezzo fa, prima della svolta abolizionista attuata con la nuova Costituzione repubblicana e democratica. Restava però un riferimento, non ancora cancellato, nell'articolo 27 della Costituzione che ammette nella formulazione vigente la pena di morte laddove sia prevista dai codici militari,

Signor Presidente, perfettamente conscio della necessità

*(UDC)*. Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC voterà convintamente a favore di questo provvedimento. Il rifiuto della pena di morte si radica nella coscienza del popolo italiano dopo la tragedia sanguinosa della Seconda guerra mondiale. Troppo abbiamo subito la violenza ed il sangue; troppo abbiamo subito una guerra provocata da due opposti totalitarismi, quello nazi-fascista e quello comunista. ha inciso sulle nostre coscienze, sulle carni vive dei popoli europei. Da lì nasce il rifiuto della pena di morte. Nel dramma dei totalitarismi i popoli europei hanno riscoperto, nella visione cristiana della persona umana e della sua dignità trascendente e intangibile, l'unico punto di riferimento morale al quale orientare le proprie azioni. Per questi motivi, il disegno di legge che oggi approviamo in via definitiva completa un grande percorso ideale che sta alla base della coscienza del popolo italiano. Sarei ipocrita se in questo momento non ricordassi però che, se nessuno deve toccare Caino, non abbiamo il diritto di dimenticarci di Abele. Bandire la pena di morte significa dire che uno Stato degno di questo nome deve tutelare la sicurezza dei cittadini, senza usare la pena di morte con modi più civili e più efficaci. Ma negare la pena di morte significa assumere questo obbligo con convinzione e decisione ancora maggiori. Non posso non ricordare la stridente contraddizione che esiste tra la legge che ci apprestiamo ad approvare ed il tentativo di introdurre nell'ordinamento repubblicano l'eutanasia, cioè la soppressione della vita innocente, come non posso non dire come questo si lega al dramma sanguinoso dell'aborto che permane come una vergogna all'interno dei Paesi occidentali.

Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, non è né un caso né una cosa banale che questo provvedimento giunga in un'Aula del nostro Paese perché, come è noto a tutti, il primo Stato al mondo che abolì la pena di morte fu il Granducato di Toscana, segno della presenza di una cultura illuminista che reggeva quegli ordinamenti, che pure non erano italiani ma degli Asburgo-Lorena. questa tradizione fa da corona anche la ricca produzione giuridica napoletana che, già dal tempo della rivoluzione giacobina, illustrò

a dimostrazione che anche in un periodo in cui l'Italia era ancora divisa in molti Stati, tanto che Metternich poteva definirla un'espressione geografica e non politica, esisteva una cultura comune, soprattutto sui fondamenti giuridici. Questo mi sembra un elemento molto importante da ricordare per dare a questo voto un respiro. Abbiamo bisogno, in momenti di particolari meschinità, pettegolezzi, rivalse, di temi che ci obbligano a fare i conti con la nostra grande storia per valutarla non in modo nazionalistico o trionfalistico, ma nei suoi valori fondativi reali, nel suo spessore. Rimane vero quello che già Beccaria dimostrò: la pena di morte non rimedia il delitto né lo riduce. Tutti gli Stati dell'Unione americana, in cui vige la pena di morte, non hanno fatto registrare una qualsiasi riduzione dei crimini. Questa pena è irreversibile e non consente di mettere riparo ad un qualsiasi errore giudiziario e, soprattutto, secondo noi che appoggiamo con grande vigore questo testo, incrudelisce anche le relazioni. Non è vero che la sicurezza dei cittadini poggia sull'aumento della paura. La paura e la fame, come dice un vecchio proverbio popolare, sono cattive e non buone consigliere. E' molto più importante stabilire un'autorità benevola e significativa dello Stato, fondata su un diritto pieno di civiltà, che abbia insieme l'idea della giustizia ma anche della clemenza, l'idea della sua forza ma anche del suo limite. L'onnipotenza del diritto è sicuramente una cosa che non si può sostenere, è sbagliata, induce altre onnipotenze che poi diventano, per la verità, possibili Trovo che ci sia una fondamentale distinzione tra la tradizione del diritto che chiamiamo romano e quella del diritto che chiamiamo anglosassone proprio su questo punto. che nell'ordinamento degli Stati Uniti i parenti delle vittime abbiano il diritto di assistere all'esecuzione della pena di morte significa che lo Stato si considera solo esecutore della vendetta privata e la fa diventare un po' più civile, nel presupposto che la pena

il diritto perde la sua caratteristica di terzietà, di momento di grande equilibrio etico tra un'infrazione e un riparo, per quanto possibile, e diventa l'esecuzione di una vendetta.

un bell'esempio di conoscenza equilibrata e razionale della nostra grande tradizione e diamo anche un senso alla voglia che abbiamo di convivenza civile tra noi, retta dal diritto e anche dalla solidarietà, dalla

Chi vi parla è contrario alla pena di morte, in quanto la ritiene non soltanto disumana ma anche inutile. È dimostrato che non è un deterrente che possa servire a diminuire i delitti, né a distogliere chi commette i reati dal compierli. Vorrei però sottolineare alcuni aspetti che francamente non mi piacciono di questo dibattito, che si è dipanato per qualche mese, così come vuole la Costituzione. Intanto, perché, di fatto, è privo di significato, se non di un significato simbolico. Ricordo che la pena di morte nel nostro Paese è stata già abolita, non valeva per i civili e proprio recentemente è stata abolita anche la

in realtà ha l'odore di una sorta di *fumus* propagandistico. Anche in questa Aula è riecheggiata la rivendicazione che all'ONU si parla della pena di morte perché l'Italia ha appunto imposto questo ordine del giorno. Se così fosse, e così forse è, si tratta dell'unico merito che questo disgraziatissimo Esecutivo, che sta rovinando questo disgraziatissimo Paese, può vantare in questo anno e mezzo di Governo che ha scontentato tutti gli italiani. Non mi sembra che un tema così importante si debba prestare a questioni di natura propagandistica;

dei cittadini). Ricordo appunto la pena di morte che noi, per ignavia e per negligenza, infliggiamo ai tanti Abele che ci sono anche nel nostro Paese, lasciando liberi i criminali, non garantendo la sicurezza, e facendo sì, attraverso la nostra mancata azione legislativa e anche amministrativa, che anche Caino debba essere esente dalla pena di morte. Ricordo poi il tema dell'eutanasia, che credo sia sinistro ma che continua ad aleggiare anche in queste Aule. Bene, ricordiamoci, quando questi temi magari verranno affrontati anche in Aula, che oggi abbiamo votato contro la pena di morte nella nostra Costituzione. Il tema è talmente delicato che la Lega Nord lascia libertà di coscienza

mi impongono di fare una brevissima valutazione. Starei molto attento a determinare un meccanismo culturale in base al quale si crea un automatismo tra totalitarismi e pena di morte,

la riflessione di chi tende a distinguere tra Europa ed Occidente e a non far coincidere il modello occidentale con quello europeo. Pertanto, alcune affermazioni che appaiono rigorose dal punto di vista filosofico, storico e culturale, in realtà, aprono qualche crepa nel dibattito e nella riflessione politica e culturale. Vorrei aggiungere un'altra considerazione:

ma credo che il Parlamento adesso si debba assumere un'altra responsabilità. Abolita la pena di morte, anche nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, resta ancora nel nostro Paese chi la pena di morte quotidianamente la infligge e sono coloro i quali, impuniti, espressione della criminalità di questo Paese, continuano ad imporla, soprattutto in alcune aree

Buttiglione e Castelli: ricordiamoci di Abele e non solo di Caino.

che cancella definitivamente dal nostro ordinamento la pena di morte. Credo che sia un risultato ampiamente condivisibile, una scelta alta che ha un profondo valore morale e che condividiamo fino in fondo. Pertanto, fin d'ora, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. Credo che questo risultato debba essere condiviso sotto il profilo

la pena di morte e in modo subdolo e violento. Penso che il senatore Silvestri, quando attacca Israele, dimentichi le parole del Presidente iraniano, il quale fino a ieri, in in terra americana, ha negato l'Olocausto. Vorrei vedere il senatore Silvestri impegnato a difendere in modo identico il diritto dello Stato di Israele e dei suoi cittadini di esistere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, questo disegno di legge costituzionale torna in Aula al Senato proprio nei giorni in cui si apre la 62a Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella quale l'Unione Europea, con una voce sola, grazie ad un impegno particolare del nostro Governo, ma anche dell'Italia intera, insieme ad altri Paesi, in rappresentanza di tutti i Continenti, chiederà di approvare una moratoria universale contro la pena di morte. Questa azione comune ha il sostegno dell'opinione pubblica e trova la massima condivisione politica in Italia. Oggi la potremo testimoniare con questo voto in Aula e dire che siamo tutti convinti della sacralità della vita umana anche dinanzi ad una legittima pretesa dello Stato di vedere puniti i colpevoli di gravi reati che oggi, secondo l'articolo 27 della nostra Costituzione, potrebbero essere perseguiti, appunto, con la pena di morte in circostanza di guerre e per violazione di leggi militari. L'etica dello Stato moderno non può prescindere dal rispetto dei valori per i quali pretende il rispetto da parte dei propri cittadini, né può confondersi l'argomento con l'etica dei privati al rispetto della vita che lo Stato ha il dovere di promuovere. La differenza si coglie in tutta la sua interezza riflettendo proprio sul testo legislativo in esame e sulle sue conseguenze: l'Italia non ha potuto ratificare il XIII Protocollo allegato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, per il quale non è consentita alcuna deroga o riserva. Infatti, anche se nel 1994 con la legge n. 589 abbiamo abolito la pena di morte nel codice penale militare di guerra, la residua previsione costituzionale dell'articolo 27 consentirebbe una sua reintroduzione in ogni momento. dunque, ha sottoscritto il Protocollo, ma non l'ha potuto ratificare. Approvando questo disegno di legge, diamo un chiaro senso politico alla nostra decisione di aborrire la soppressione della vita umana in qualsiasi circostanza per una giusta intransigenza verso l'eticità dei comportamenti dello Stato, ma anche per un chiaro sostegno all'azione del Paese verso l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo provvediamo anche a superare un vincolo giuridico che ci impedisce di adempiere ad un Trattato internazionale come la Convenzione sui diritti dell'uomo e, segnatamente, il XIII Protocollo, che certamente qualifica il livello di civiltà dei Paesi che l'hanno sottoscritto e ratificato. Pertanto, non possiamo che auspicare l'immediata e definitiva approvazione del disegno di legge al nostro esame con il più ampio consenso di quest'Aula che già si preannunzia. A questo consenso daremo il nostro contributo. L'Ulivo garantirà il voto favorevole sperando di contribuire, insieme agli altri Gruppi politici presenti in quest'Aula, a sostenere un movimento che vada oltre i confini del nostro Paese capace di limitare le tante atrocità che ancora si consumano in troppe parti del mondo con la soppressione della vita umana per una decisione legittima, ma sempre ingiusta degli Stati che ancora lo consentono. *(Applausi

di una penalizzazione che contrasta con i principi del nostro ordinamento e con il valore della vita. Sottolineiamo anche noi, come qualche oratore ha già fatto, il valore della vita evocato nel corso della discussione,

mondiale che miri al superamento della pena di morte anche in quei Paesi dove questo strumento giuridico viene ancora praticato. Presidente, personalmente sono contrario alla pena di morte, ma ritengo che in questo caso stiamo discutendo un problema particolare, cioè la pena di morte in tempo di guerra. Per ragioni professionali, conosco la drammaticità di determinati momenti e so che la storia del nostro Paese e la storia della libertà e della democrazia sarebbero state diverse se non ci fosse stato questo strumento. Certo, la guerra è cambiata e cambia nel tempo e oggi non ci sono più quelle situazioni drammatiche createsi al tempo della Prima e della Seconda guerra mondiale, ma mi pare che questo aspetto nel dibattito non sia stato tenuto nel debito conto. Non ho sentito quella drammaticità che avrei auspicato e non ho sentito argomenti che mi hanno del tutto convinto. Per questo motivo, ritengo un dovere annunziare che non prenderò parte al voto. So perfettamente che questa posizione è fortemente impopolare e anche fortemente minoritaria persino nel mio Gruppo, ma credo che in certi momenti sia necessario, per i senatori in quest'Aula, non nascondersi dietro un ipocrita «non spingere il pulsante», ma dire le ragioni delle proprie perplessità e del proprio dissenso.

Tutti confidano in lei, senatore Silvestri. Non voglio dilungarmi perché ho troppo rispetto per quest'Aula e per il popolo che rappresentiamo per pensare che qualcuno possa essere a favore della tortura, essendo il il rispetto della persona umana e il rispetto dell'intangibilità del corpo e della propria esistenza uno dei dati fondanti in base a cui anche questa Assemblea

sempre. Anche quando discutiamo di immigrazione e di rientro degli immigrati in alcuni Paesi, dobbiamo valutare attentamente se lì non esista anche la tortura per non rischiare di rimandare persone in uno Stato che non rispetta gli *standard* minimi di civiltà.

registriamo casi internazionali in cui alcune potenze che vietano la tortura e gli interrogatori pesanti sul proprio territorio usano altri Stati (tra l'altro, Stati

chiaramente, come Gruppo, siamo convintamente a favore dell'introduzione del reato di tortura. La tortura, così come il genocidio, è considerata un crimine contro l'umanità dal diritto internazionale. La proibizione della tortura e di altre forme di trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti costituisce l'oggetto di molteplici convenzioni internazionali ratificate anche dal nostro Paese. Sebbene i metodi di tortura praticati nel mondo si siano andati raffinando, non è difficile trovare un accordo su cosa debba intendersi per tortura. Sul punto ci soccorrono l'esperienza storica, gli scritti dei grandi illuministi (citati anche dal relatore - oggi assente, il senatore Buccico - in Commissione: Verri, Beccaria, Voltaire, Manzoni), i racconti dei dissidenti politici che l'hanno subita. Ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (ad esempio, quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio usate nell'Irlanda del Nord o in Spagna), e il rapporto della Commissione europea dei diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli. Ci è quindi sembrato evidente che la tortura fosse qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni, oppure per umiliarla, punirla o intimidirla. Nella tortura la disumanità è deliberata: una persona compie volontariamente contro un'altra atti che non solo feriscono quest'ultima nel corpo o nell'anima, ma ne offendono la dignità umana. Nella tortura c'è, insomma, «l'intenzione di umiliare, offendere e degradare l'altro essere umano, di ridurlo a cosa», come si esprimeva Antonio Cassese nelle sue memorie di presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti. degradanti. La Convenzione delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, all'articolo 1 definisce il crimine della tortura come: «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito». All'articolo 4 si prevede che ogni Stato consideri tali atti quali trasgressioni nei confronti del proprio diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura. Nasce, quindi, un obbligo giuridico internazionale che deve essere rapidamente adempiuto dal nostro Paese, con l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitato sia dal Comitato sui diritti umani istituito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato ai sensi della legge n. 881 del 1977, sia dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 1989, n. 7, il quale, nell'esame dei rapporti periodici sull'Italia, ha sottolineato più volte come fosse necessario supplire a tale lacuna normativa. La proibizione della tortura è prevista all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dal nostro Paese.

compimento dell'approvazione di questo disegno di legge, una mostra che ricordi quanto è accaduto ad Abu Ghraib. Vorrei ricordare che il disegno di legge non c'entra assolutamente nulla con Abu Ghraib, perché quanto è accaduto lì è stata una violazione delle leggi dell'Iraq e degli Stati Uniti d'America che proibiscono la tortura. La tortura naturalmente - detto per inciso - è proibita anche in Italia; sarebbe già stata proibita prima, qui se ne fa un reato specifico da punire in modo specifico, come è giusto e come tutti sosterremo con il nostro voto a favore, ma far passare Abu Ghraib come un caso di tortura legale è veramente un falso. Se vogliamo fare le mostre delle torture legali, cioè la tortura fatta per ordine e con il consenso dello Stato,

Paesi del mondo (parliamo delle amputazioni fatte per l'applicazione di certe leggi che sappiamo). Questa è una cosa che forse potremmo pensare di fare, ma far passare Abu Ghraib come un caso di tortura legale, che una legge avrebbe impedito, è assolutamente un falso. Chi ha perpetrato quanto è successo ad Abu Ghraib è stato perseguito dalla giustizia del suo Paese ed è stato condannato secondo giustizia e con i processi, con le dovute garanzie; sono stati abusi puniti dalle autorità che ne avevano la competenza. Ben altri sono gli episodi che vanno ricordati; non pensiamo che la tortura perpetrata dallo Stato, con il consenso dello Stato in certi Paesi sia sia cosa che appartiene al passato; purtroppo, succede ancora oggi. Però, senatore Silvestri, questo non succede in Iraq e tanto meno negli Stati Uniti d'America; succede in altri posti e mi meraviglio che lei, che è sensibile ai diritti umani, abbia alimentato questo sospetto. Ben altro è quello che succede, sono altri i Paesi e di questo credo dovremo occuparci in altra sede, non in questa. Signor Presidente, la legge è politicamente corretta, quindi questo ammasso del politicamente corretto ormai troverà il consenso di tutti, per carità. Giustamente è politicamente corretto essere contro la tortura. Vorrei sapere chi è a favore della tortura nel nostro Paese; vorrei che qualcuno mi dicesse dove, quando e come viene perpetrata la tortura nel nostro Paese.

psichiche o condiziona il comportamento, oppure discrimina è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Ora, il concetto di sofferenza psichica è abbastanza largo; largo; chiunque eserciti il principio dell'autorità può essere accusato di infliggere sofferenza psichica. In particolare, sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio anche gli insegnanti di scuola pubblica. L'insegnante di scuola pubblica che si presenta in una classe e dice «se non salta fuori il colpevole di questo atto siete tutti sospesi; domani salti fuori il responsabile», è accusato di tortura.

il pilota d'aereo che dica «state seduti altrimenti precipitiamo» provoca una sofferenza psichica. Nella maglia del politicamente corretto tutti possono essere accusati. Il politicamente corretto ormai è diventato la nuova inquisizione, la Santa Inquisizione.

in base alla casacca che si indossa, tutto è consentito. A Cuba tutto è consentito: fucilano o mettono in galera gli omosessuali e c'è ancora qualche Ministro che si commuove

nei *gulag* qualcuno c'è stato. Anche questa potrebbe essere un'induzione di sofferenza psichica? Vi è altresì un'altra categoria, molto più debole, e la tortura è qualcosa di ignobile se praticata verso una persona debole.

da sindrome di Down sì. Questa è un'ipocrisia; se si tutela la vita, la si tutela sempre. Se lo Stato non può disporre della libertà delle persone e non può essere coercitivo, non può disporre e fare il processo sommario dell'embrione, insieme con il vostro Ministro o con tutti gli sproloquiatori, a partire dal ministro Bonino o altri. Quella non è libertà, bensì omicidio ed è molto più grave

la discussione dei disegni di legge relativi al rendiconto e all'assestamento del bilancio dello Stato avrà luogo in apertura della seduta pomeridiana di domani.